che riguarda il motivo per il quale il legislatore ha previsto l'Agenzia di cui lei ha fatto menzione e quali sono le funzioni che le ha delegato:

che nella volontà del legislatore dovrebbe rafforzare la parte datoriale pubblica nelle trattative con i sindacati al fine di garantire la compatibilità economico-finanziaria dei rinnovi dei contratti dei lavoratori pubblici con gli obiettivi e l'equilibrio del bilancio. Faccio questa premessa perché alla luce di essa è più facile intendere l'importanza del rapporto trimestrale che l'ARAN ha il compito di stilare e di comunicare al Parlamento, al Governo e ai Comitati di settore. Non vorrei, visto che su questa materia sono più volte tornato ad interrogare il Governo e ad approfittare della cortesia del sottosegretario Scanu, che questa richiesta venga scambiata come una gentile concessione che l'ARAN deve all'opposizione o a un senatore particolarmente zelante. Il rapporto trimestrale è di importanza fondamentale perché consente al Parlamento di svolgere le sue funzioni di controllo sull'attività negoziale del Governo e di valutare questa attività e, più in generale, è di fondamentale importanza per comprendere un settore

necessari e significativi confronti con l'andamento delle retribuzioni nell'ambito privato e deve prevedere per forza di cose una specificazione per i vari comparti di contrattazione; solo così diventa un documento significativo e importante. E questo, torno a sottolinearlo, è previsto da una legge dello Stato. Ebbene, la vicenda di detto rapporto trimestrale è quanto mai singolare. Oggi abbiamo assistito, in questo Parlamento, all'andata in onda di una maggioranza introvabile e potremmo parafrasare la stessa espressione per questo rapporto: il rapporto introvabile. il rapporto trimestrale non è trimestrale, non viene pubblicato nei momenti in cui se ne sente effettivamente la necessità, non riporta i dati che sarebbe auspicabile trovare: salvo che per un periodo estremamente ristretto, nel corso della prima parte dell'anno 2006, questo rapporto è sempre lacunoso. Cosa è accaduto ultimamente (e su questo verte la interpellanza al Governo)? È accaduto che il rapporto non è stato pubblicato alla scadenza del trimestre; lo abbiamo visto apparire sul sito dell'ARAN solamente nel mese di giugno; i suoi dati erano aggiornati all'aprile dunque erano aggiornati ad un momento nel quale non erano più ufficiali, e fino al 25 luglio, ultimo giorno nel quale ho interrogato gli uffici del Senato, esso non era stato ancora trasmesso alle Camere. Devo dire che questa situazione, oltre ad essere illegittima, è anche offensiva per il Parlamento, perché un rapporto per quanto invecchiato e in grande parte inutile, nel momento in cui viene pubblicato sul sito dell'Agenzia, sarebbe buona creanza che fosse ricevuto anche dalle Camere, cui per legge è innanzitutto destinato.

ma soprattutto non riportava - e questo è stato notato persino in sede europea ed evidenziato come rilievo - i necessari raffronti con l'andamento delle retribuzioni nel settore privato. Questo dato è importante e fondamentale non solamente per comprendere se all'interno di questo settore vi è un equilibrio, ma anche per capire quale tipo di correzione è nel caso necessario

dall'ARAN, che è l'Agenzia che - lo ripeto ancora una volta - per legge è tenuta a fornirli, è possibile talvolta rintracciarli all'interno dei bollettini dell'ISTAT in maniera più precisa, più dettagliata e più aggiornata. Questo è il motivo per il quale una delle richieste avanzate al Governo è quella di prendere atto di una realtà - e noi l'abbiamo fatto proponendo un disegno di legge in materia

più al riparo da pressioni di tipo sindacale. Questo al fine di dare la possibilità ai parlamentari di svolgere quell'attività di controllo che, attraverso ritardi programmati e in qualche modo

in via preliminare, intendo ricordare che, come ho già avuto modo di chiarire il 12 aprile scorso nel rispondere ad una interrogazione su analogo oggetto, il comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è stato integralmente ricostituito, con le modalità e sulla base delle designazioni acquisite ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006. Fino a tale data, quindi, a causa dell'assetto incompleto il comitato non ha potuto assicurare il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia, tra le quali - come rilevato dal senatore interpellante anche la predisposizione del rapporto trimestrale sulle retribuzioni del pubblico impiego. In particolare, in merito alla lamentata inadempienza relativa alla puntuale pubblicazione del rapporto trimestrale risulta di tutta evidenza che il ritardo è stato dovuto alla circostanza che la piena ed effettiva operatività dell'ARAN è stata ripristinata, per le ragioni sopra ricordate, soltanto a partire dal gennaio 2006. Del resto, la soluzione di continuità stigmatizzata dall'interpellante, determinatasi a causa dell'avvicendamento delle nomine apicali dell'Agenzia negli ultimi mesi del 2006, trova riscontro anche in precedenti esperienze, così come dettagliatamente documentato nell'elenco dei rapporti consultabile sul sito *web* dell'Agenzia. Da tale elenco è infatti possibile evincere che la cadenza trimestrale di pubblicazione dei rapporti è stata rispettata solo fino al 1999. Successivamente, la pubblicazione dei rapporti ha sempre avuto cadenza semestrale. L'interpellanza presentata il 25 luglio scorso sostiene inoltre che fino a tale data il rapporto non sia stato formalmente trasmesso al Parlamento e che, invece, sia stato irritualmente reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia. Al riguardo è utile ricordare che soltanto le prime edizioni del rapporto, dal 1998 fino a parte dell'anno 2000, sono state trasmesse in formato cartaceo alle competenti Commissioni parlamentari. L'avvento di Internet, infatti, e proprio l'esigenza di tempestività a cui si appella il senatore Quagliariello hanno consigliato, per gli anni successivi, di avvalersi dello strumento informatico, tecnicamente più efficace e tale da assicurare una più ampia e capillare diffusione. Peraltro, l'adempimento formale della trasmissione del rapporto in formato cartaceo è stato in ogni caso rispettato, predisponendone la consegna ai 200 destinatari istituzionali, tra i quali i Presidenti di tutte le Commissioni parlamentari ed i responsabili del Servizio bilancio di Camera e Senato. Infine, in merito alle omissioni conoscitive lamentate dal senatore interpellante, relative alla mancata considerazione ed analisi nell'ambito del rapporto dei dati sulle retribuzioni di fatto nel 2006, nonché di quelli riferiti al settore privato, si precisa innanzitutto che il rapporto, in quanto redatto sulla base delle informazioni disponibili al 30 aprile 2007, non ha potuto ovviamente tenere conto dei dati riferiti al 2006 e forniti dall'ISTAT e dalla Banca centrale europea nella prima metà del successivo mese di giugno. Il rapporto è stato quindi diffuso contemporaneamente alla messa a disposizione delle suddette informazioni. Tali elementi pertanto non potevano formare oggetto dell'approfondito lavoro di analisi, valutazione e sintesi garantito dal rapporto ARAN. Peraltro, si anticipa che gli atti relativi al 2006, lungi dall'essere trascurati, costituiscono invece il punto centrale del rapporto attualmente in preparazione, che comprenderà, insieme alle stime di contabilità nazionale, le valutazioni condotte sulla base del campione ARAN per i principali comparti delle amministrazioni non statali. Il rapporto in questione, in fase di avanzata realizzazione, verrà reso disponibile entro la fine del corrente mese di settembre. Va inoltre chiarito che il rapporto del maggio 2007 costituisce il completamento della precedente edizione dell'agosto 2006. In quest'ultimo erano state infatti presentate le risultanze del campione ARAN con riferimento ad enti locali ed enti sanitari, inquadrando i relativi dati nel contesto più generale delle amministrazioni pubbliche e raffrontandoli inoltre con il segmento dell'industria in senso stretto che, tradizionalmente, rappresenta il settore privato. L'ultima edizione del rapporto (quella di maggio 2007) fornisce, quindi, il completamento dell'analisi delle amministrazioni non statali, utilizzando risultanze aggiornate al 2005, in relazione ai comparti di contrattazione collettiva di enti pubblici non economici, università e ricerca. Da quanto detto risulta di tutta evidenza che il rapporto trimestrale frutto di un costante impegno di raccolta, elaborazione e analisi di dati - rappresenta una essenziale fonte di informazioni sulle retribuzioni del settore pubblico ed uno strumento di conoscenza utile alla programmazione delle politiche retributive pubbliche. Strumento che, stante la sua elevata connotazione tecnica, non può che essere fornito da un organismo, quale, appunto, l'ARAN, deputato per sua natura a curare attività di analisi fortemente specializzate e tale, quindi, da garantire risultati di elevato livello qualitativo. Si tratta, infatti, di vere e proprie elaborazioni a carattere non esclusivamente statistico, che, pertanto, non possono essere efficacemente fornite da organismi aventi natura diversa (è il caso dell'ISTAT). Al riguardo non va dimenticato che, proprio attraverso il monitoraggio dell'andamento della contrattazione collettiva - e, in particolare, delle retribuzioni -l'ARAN è in grado di apportare un ausilio fondamentale alla realizzazione di efficaci processi di innovazione e riqualificazione nelle pubbliche amministrazioni.

molto scontento e insoddisfatto della sua risposta. Ho fatto per vent'anni il professore universitario e sono abituato a considerare il tempo elasticamente: si dice che per il professore universitario l'anno dura sei mesi, il mese 20 giorni, il giorno sei ore e l'ora 50 minuti; però, da questo al fare il gioco delle tre carte ne passa e devo dire che rivaluto a questo punto la concezione del tempo dei miei colleghi rispetto a quella che ci ha proposto. Questo perché innanzitutto, il 25 innanzitutto, il 25 luglio, interpellati gli Uffici del Senato, mi è stato detto che il rapporto non era stato comunicato; certo che lo si può vedere sul sito Internet, ma ritengo che una comunicazione ufficiale, di cui lei dà conto, ma non si sa quando è avvenuta, sia comunque necessaria perché il parlamentare possa esser certo che quello che vede sul sito sia ufficiale e conforme a quello che è stato comunicato per le vie brevi. Credo che l'informatica non sia ancora arrivata al punto di stravolgere le prassi istituzionali. In secondo luogo, mi permetterei di rileggere quello che lei ha detto alla luce di una concezione del tempo più veritiera, diciamo meno elastica. Come lei ci ha detto, prima di questo, l'ultimo rapporto trimestrale risale all'agosto 2006; da allora avremmo dovuto vederne pubblicato uno per il novembre successivo, cioè tre mesi dopo, ma in quel periodo il Governo era impegnato a sostituire i vertici ARAN, quindi è ipotizzabile che, in assenza dei propri vertici, l'ARAN abbia pensato di rinviare la pubblicazione, arrivando così al semestre successivo. Ma neanche nel febbraio 2007 abbiamo avuto notizie dell'ormai famigerato rapporto trimestrale ARAN; abbiamo dovuto attendere lo scorso mese di giugno per avere notizie ufficiose come lei ci ha detto - sul rapporto trimestrale, poiché lo abbiamo rinvenuto sulle pagine Internet dell'Agenzia. Con una pratica poco decorosa, il rapporto veniva datato maggio 2007. Questo ovviamente non per un vezzo, ma per giustificare l'assenza - e lei ce lo ha spiegato - dei dati elaborati dall'ISTAT e resi pubblici i primissimi giorni di giugno, cioè il 5 giugno, per esattezza, che avrebbero consentito all'ARAN di elaborare l'andamento delle retribuzioni di fatto a tutto il 2006; dati che - come le risultanze dimostrano - hanno evidenziato come il divario tra la crescita delle retribuzioni del settore pubblico rispetto a quelle del settore privato privato sia ulteriormente aumentato. Non è un caso che il bollettino della Banca centrale europea del giugno 2007 abbia denunciato l'anomalo andamento delle retribuzioni nel nostro Paese tra settore pubblico e settore privato, denunciando come l'aumento della retribuzione *pro capite* nel settore pubblico (più 36 per cento) sia stato negli ultimi anni più che doppio rispetto ai tassi di incremento delle retribuzioni *pro capite* nel settore privato (14, del tutto fuori linea rispetto alla media dei Paesi europei. Ovviamente, non bisogna essere degli economisti per capire che siffatta tendenza è dirompente per il sindacato del pubblico impiego. Come giustificare altrimenti - e concludo, Presidente - le proprie richieste davanti al Governo, davanti a dati così eclatanti? Il dubbio vero, però, è che il Governo sia connivente con la strategia del sindacato e che questa sia la ragione effettiva dei ritardi, delle omissioni e dei momenti puntuali, nei quali i rapporti sono apparsi. D'altra parte, se il tempo è a geometria variabile ma non è proprio un'opinione, se proprio non vogliamo applicare il massimo del relativismo al tempo, gli ultimi dati del rapporto ARAN - Agenzia pienamente insediata che ha impiegato sei mesi, secondo la sua

Restiamo in attesa, legati ad una promessa di cui vedremo le sorti a fine settembre. Speriamo che l'elasticità del tempo dell'Agenzia ARAN non venga del tutto meno, ma quanto meno si riduca.

Signor Presidente, il completamento degli intereventi di risanamento acustico lungo la strada statale n. 47 "della Valsugana", già iniziato in alcuni tratti, è stato oggetto, a seguito delle numerose sollecitazioni pervenute da parte delle istituzioni e delle popolazioni locali, di particolare attenzione da parte di ANAS. La società stradale ha pertanto inserito l'intervento in questione tra le priorità del piano di risanamento acustico della rete stradale nazionale e, da ultimo, nel piano di manutenzione straordinaria come opera di nuova realizzazione nell'ambito del contratto di programma firmato con il Ministero delle infrastrutture lo scorso 28 giugno. Il Ministero si impegna pertanto a far sì che la realizzazione delle opere di mitigazione acustica nel tratto della strada Valsugana in questione sia considerato dalla società stradale uno dei punti cui dare priorità nell'ambito delle attuali disponibilità finanziarie.

l'ANAS e, quindi, il Governo hanno capito la necessità di questo intervento e si siano impegnati a realizzarlo in tempi brevi; riserva perché nella sua risposta non sono indicate né date né tempi precisi di realizzazione, per cui

della superstrada Valsugana queste barriere fonoassorbenti sono state realizzate fin da quattro anni fa, mentre sull'altro lato, tra l'altro il più popoloso, questo intervento non ha avuto luogo fino ad oggi.

fino ad oggi lettera morta e che solo ora trovano accoglimento, almeno stando alle sue parole, per quanto riguarda la realizzazione di questo intervento. Quindi, sotto un profilo di politica generale, è sconfortante verificare che opere

in esito alla richiesta di informazioni per la risposta all'interrogazione in oggetto, con la quale sono stati posti alcuni quesiti in ordine, tra l'altro, alla conferenza di servizi tenutasi presso il Ministero delle infrastrutture ai fini della localizzazione dell'autostrada A9, tratta Lainate-Como, si fa presente quanto segue. La realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9 risulta inserita tra le priorità infrastrutturali che interessano il territorio della Regione Lombardia, all'interno de! documento "Infrastrutture prioritarie" recepito nell'"allegato Infrastrutture" al nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria. Per quanto attiene al dissenso espresso dal Comune di Uboldo e con specifico riferimento, quindi, a quanto richiesto dal senatore interrogante in ordine alle misure che si intendono adottare ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241), corre l'obbligo di precisare che la conferenza di servizi per l'accertamento di conformità urbanistica delle opere di interesse statale è disciplinata non già dalle norme recate dalla legge n. 241 del 1990, bensì dalla speciale normativa dettata dal decreto del ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale). In virtù del richiamo operato dall'articolo 4 del citato decreto n. 383, le ipotesi di mancato perfezionamento dell'intesa Stato-Regione ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica, sono regolate, pertanto, dall'articolo 81, comma 4, del n. 616, in base al quale si provvede, in, tali casi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Ciò posto, si fa presente che, in data 20 luglio ultimo scorso, si è tenuta, presso il competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture, una riunione tecnica con il nuovo sindaco del Comune di Uboldo, a seguito della quale, anche sulla base anche sulla base di quanto dallo stesso previamente concordato con la Regione interessata, si è convenuto di riaprire la conferenza di servizi, al fine di pervenire, in tempi rapidi, ad una soluzione condivisa sulle questioni poste dal Comune dissenziente. La riunione della Conferenza di servizi si terrà nel prossimo mese di ottobre, in attesa della definizione dei ricorsi proposti avverso i risultati elettorali che hanno interessato il Comune di Uboldo successivamente alla pronuncia del TAR fissata per il 9 ottobre. La questione sollevata potrà pertanto essere risolta attraverso la revisione del parere reso in conferenza di servizi dal Comune di Uboldo, con conseguente raggiungimento dell'intesa Stato-Regione, ovvero mediante l'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il presidente della conferenza medesima potrà rimettere gli atti ai sensi dell'articolo 81 del decreto

Massimo rispetto per il Comune di Uboldo, ma massimo rispetto anche per gli altri Comuni - e sono veramente tanti - che, già da tempo, hanno sottoscritto in Conferenza di servizi ogni tipo di accordo tanto di rispetto anche a quei milioni di automobilisti e di autotrasportatori costretti sulla tratta autostradale A9 a code snervanti in condizioni, molto spesso, prive prive di sicurezza. Noi attendiamo sinceramente l'opera. Mi auguro che il riferimento ai tempi rapidi contenuto nella sua risposta sia reale perché non voglio essere polemico, ma la valutazione d'impatto ambientale, a causa del ritardato parere espresso dai ministri Pecoraro Scanio e Rutelli, ha allungato l'*iter* di questa pratica di oltre un anno. anno. Non vorremmo che, approfittando dell'ennesima Conferenza di servizio, qualche altro Comune, onorevole Sottosegretario, chiedesse ulteriori modifiche al progetto. Ciò sarebbe veramente disastroso per la cantierizzazione dell'opera.

anche con il precedente Governo, in questi anni - però, altre opere considerate prioritarie per la Lombardia, come la Pedemontana o alcuni interventi sulla strada statale Regina del lago di Como, sono ancora ferme al palo. Massima fiducia, quindi, nell'amico sottosegretario Casillo, ma la nostra gente è veramente stanca. L'economia e il turismo risentono molto di questo *gap* infrastrutturale. La Società Autostrade prevede ufficialmente la consegna dell'opera finita per il 2009; lei pensi che la prima previsione risaliva al 2007. Faccio appello a lei, onorevole Sottosegretario, e al Governo affinché la burocrazia, dal momento che questa infrastruttura è finanziata e anche progettata, non rallenti ulteriormente la consegna dell'opera finita, così come previsto anche da Società Autostrade. Quindi, attendiamo con molta ansia la Conferenza dei servizi di ottobre e poi, finalmente, il progetto definitivo e la cantierizzazione.

Come richiesto nella interrogazione del senatore Battaglia, abbiamo avviato un'ispezione dalla quale si è evidenziata la sostanziale veridicità (con qualche particolare differente) della segnalazione che era stata effettuata. Pertanto, vista l'anomalia e la irregolarità di una situazione di questo tipo, non conforme peraltro ai principi contenuti nella circolare n. 74 del 21 dicembre 2006 (quella relativa all'iscrizione e alla modalità di costituzione della classe), abbiamo provveduto affinché fossero date disposizioni per evitare che l'andamento dell'anno scolastico, nel quale le classi non potevano più essere suddivise, arrecasse pregiudizio per i bambini di quella classe. Sono state quindi create attività didattiche interclasse, è stato

quello dello scorso anno; si trattava di un dirigente reggente, il che significa che aveva due diverse scuole e anche questo può aver ingenerato qualche difficoltà nel seguire la vicenda. Da quel che ci risulta, quest'anno nella scuola non si sono verificate situazioni di quel tipo. comunque, nuovamente un'ispezione specifica all'interno della scuola stessa. Colgo positivamente, e confermo che stiamo vigilando, l'osservazione contenuta nell'interrogazione di

ricordo al senatore interrogante che la legge n. 1 del 2007, quella che ha innovato la normativa sugli esami di Stato, riprendendo la legge n. 425 del 1997, ha previsto che possa essere ammesso a sostenere le prove d'esame di Stato un numero di candidati esterni non superiore al 50 per cento dei candidati interni. Quindi, ogni Commissione deve essere composta per metà

precisando che tale limite è ragionevole in quanto è legato all'esigenza di evitare - cito testualmente - "che le scuole paritarie diventino sedi privilegiate di esami, a scapito della serietà dell'esame di Stato stesso", quindi una norma pienamente costituzionale. La vicenda relativa allo specifico di alcune scuole posso sintetizzarla in questo modo: le scuole conoscevano bene la normativa, hanno accolto un numero di ragazzi superiore al numero che la legge indicava, dovevano segnalare i ragazzi eccedenti perché fossero attribuiti ad altre scuole, paritarie o statali, presenti all'interno del Comune o all'interno della Provincia stessa. non hanno ottemperato a questo adempimento; si sono avute più sentenze del TAR che concedevano una sospensiva nei confronti della normativa prevista dalla legge dello Stato; il Consiglio di Stato si è pronunciato bloccando la sospensiva;, i ragazzi però - questo è importante - hanno potuto effettuare gli esami, alcuni all'interno delle scuole paritarie (questo è accaduto in Campania, dove la sospensiva ha prodotto i suoi effetti), altri all'interno delle scuole statali alle quali dovevano essere attribuiti, magari operando nella sezione suppletiva dell'esame di Stato, perché quel giorno specifico delle prove, in particolare della prima prova scritta, una parte dei ragazzi non si era presentata nelle commissioni alle quali erano stati attribuiti. Al fine di evitare questo, che è un grave disguido nei confronti della serietà dell'esame di Stato, ma soprattutto nei confronti di molti ragazzi, e ritenendo giusta - peraltro confermata dalla sentenza della Corte costituzionale - la norma che evita che vi siano commissioni composte esclusivamente di candidati esterni all'interno delle scuole paritarie, abbiamo presentato una nuova norma, che è contenuta all'interno del decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007, attualmente *in* alla Camera per la sua conversione in legge, quindi è una norma immediatamente vigente. In questo decreto-legge viene stabilito che i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede all'assegnazione dei medesimi

Signor Presidente, ringrazio la Vice ministro per la risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatto per una ragione di metodo, dal momento che l'interrogazione era del 25 giugno, quindi la tempistica della risposta era essenziale, oltre la questione di merito. Di fronte ad un'autentica emergenza com'era quella di fornire al Parlamento utili elementi conoscitivi e di valutazione rispetto alla vicenda degli esami di Stato, sarebbe stato forse opportuno portare portare a conoscenza alcuni elementi. La stessa Vice ministro ha ricordato come si sia in qualche caso verificato quello che noi richiamavamo nella interrogazione, cioè l'intervento della magistratura amministrativa rispetto alla violazione del principio di eguaglianza, per evitare, appunto, la disparità di trattamento che si è determinata tra istituti e istituti e tra Regioni e Regioni. A mio parere,

n. 147 del 7 settembre 2007. Questa è la chiara dimostrazione che si viveva in una situazione di grande incertezza.

in scuole statali di parecchie centinaia di candidati privatisti, iscritti dal mese di novembre per sostenere gli esami in scuole paritarie. Per tale motivo, il 20 giugno, davanti a numerosissime scuole paritarie della Regione, si sono svolte clamorose proteste degli studenti, che hanno richiesto perfino l'intervento delle forze dell'ordine (questo aspetto non è stato ricordato). Al fine di evitare il ripetersi per il nuovo anno di questi episodi deprecabili, deprecabili, credo sia necessario che in materia di esame dei candidati privatisti siano emanate nuove disposizioni, onde evitare in futuro dubbi e incertezze, dal momento che la normativa vigente, nei precedenti anni scolastici, è stata ripetutamente censurata dai tribunali amministrativi, a seguito di ricorsi che hanno visto il Ministero della pubblica istruzione quasi sempre soccombente. Questo è il dato sul quale

sul terreno delle riforme, soprattutto in materia scolastica, con scelte politiche che si riverberano pesantemente sui ragazzi e sul loro futuro. Credo pertanto che una più attenta riflessione,

ma non deve determinare, come ultima conseguenza, il ricorso alla magistratura. Vogliamo che la politica si riappropri di una sua centralità